Onorevoli colleghi, avverto che previ accordi intercorsi tra i Capigruppo, le dichiarazioni di voto finale sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge anticrisi sono anticipate a questa sera, alle ore 19. Pertanto, la chiama dei senatori per il voto di fiducia avrà inizio, presumibilmente, intorno alle ore 20. La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel mio intervento voglio soffermarmi essenzialmente sulla parte del decreto-legge al nostro esame che riguarda le quote latte.

attraverso lo strumento del decreto-legge, cioè in casi straordinari di necessità ed urgenza e sempre che tali provvedimenti siano convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. in spregio all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che obbliga il Governo ad emanare decreti-legge dal contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, si accetta invece che un decreto-legge sulle quote latte, che non siete riusciti a far convertire in legge in tempo utile, venga reinserito, dopo la scadenza del termine costituzionalmente previsto, in un maxiemendamento con il quale si riscrivono ben due decreti-legge il cui contenuto non è affatto omogeneo. Si tratta di una spregiudicata alchimia legislativa che, in casi analoghi, ha portato il collega costituzionalista onorevole Zaccaria a parlare di decreti Minotauro. C'è di che stupirsi. Tant'è che lo stesso presidente Fini ha esortato il Governo a mutare in sede di coordinamento il titolo del decreto-legge, sostituendo il riferimento ai settori industriali con quello più generico ai settori produttivi. Sulle quote latte, piazza di Montecitorio è stata assediata per giorni da manifestanti delle maggiori confederazioni degli agricoltori, che - lo voglio ricordare - rappresentano la stragrande maggioranza degli agricoltori onesti, sono scandalizzati da questo decreto-legge che premia l'illegalità delle frange ribelli degli splafonatori senza se e senza ma, e magari anche senza quote latte perché le hanno profumatamente vendute ad altri agricoltori che, per rispettare il loro contingente di produzione, si sono indebitati e oggi si vedono scavalcati nelle assegnazioni delle quote supplementari e calpestati nei loro diritti. Voglio ricordare che lo Stato italiano e quindi noi tutti, anche chi è allergico al latte, ha già pagato tre miliardi di euro di multe per le eccedenze produttive. Con questo decreto-legge soltanto un terzo di queste multe verrà forse restituito in comode rate trentennali ma subito, immediatamente, proprio a coloro che più hanno violato la legge e che hanno fatto lievitare tali multe, verrà assegnata gratuitamente un'adeguata quota di latte.

portato in Aula, qua al Senato, un decreto totalmente diverso rispetto a quello che avevamo pensato; non lo avete voluto accettare e qui al Senato

Effettivamente, nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera, erano state inserite nel decreto-legge alcune norme di un certo rilievo, anche grazie agli emendamenti presentati dalle opposizioni: mi riferisco all'incremento del Fondo di solidarietà nazionale e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le imprese agricole in zone svantaggiate; si tratta di due questioni che anche da parte dei banchi dell'opposizione sono state fatte presenti sin dall'inizio di questa legislatura. Queste richieste erano diventate prerogativa comune della Commissione agricoltura della Camera, a dimostrare che, quando si vuole, si può fare qualche passo importante, anche se le risorse stanziate dal Governo per il Fondo di solidarietà nazionale erano insufficienti: occorrono infatti - questo il Ministro lo sa meglio di noi più di 230 milioni di euro per coprire gli impegni già presi dai Governi per l'anno 2008 e per finanziare il 2009, pena l'impossibilità di assicurare le produzioni; questo lo avevamo chiesto anche con il decreto-legge n. 171 del 2008. Il Fondo di solidarietà nazionale è un sistema basilare a sostegno delle imprese agricole, che patiscono i condizionamenti dovuti a calamità naturali e a circostanze non prevedibili. Con rammarico e sconcerto, devo segnalare che le uniche norme positive del decreto-legge sulle quote-latte, quelle che effettivamente potevano essere lette in una chiave anticrisi per il settore agricolo del nostro Paese, sono scomparse dal testo attualmente al nostro esame, totalmente. Abbiamo quindi perso un'occasione per dare un segnale forte al settore agricolo. Il testo del decreto-legge, fondamentalmente, lo ricordo, tratta due argomenti cruciali: la rateizzazione delle multe pregresse e la suddivisione delle nuove quote assegnate al nostro Paese. Tuttavia, nell'elaborazione e nella stesura di questo decreto-legge, e nella brutta vicenda di procedura parlamentare che lo ha visto protagonista, si è fatto in modo, caro signor Ministro, anche se lei sostiene il contrario, che vi fossero allevatori di serie A e allevatori di serie B; il guaio è purtroppo che di serie B sono e rimangono quelli che hanno sempre rispettato le leggi e le regole. Dai panegirici del decreto-legge si evince che lo stesso è stato indirizzato agli eletti, cioè a quelli che hanno fatto il proprio comodo, splafonando (uso questo termine, giacché lo usa anche il nostro Ministro): insomma, quelli che hanno agito a proprio vantaggio, e non solo, ma hanno avuto anche il coraggio di aprire i famosi contenziosi. Staremo a vedere se questo decreto-legge, così com'è formulato, risolverà la questione: abbiamo dei dubbi, e credo che siano anche fondati, perché riteniamo che chi non ha rispettato le regole precedentemente - nonostante la legge n. 119 del 2003 del ministro Alemanno, che avrà sicuramente presentato punti di debolezza, ma che comunque ha offerto la possibilità agli irregolari (chiamiamoli così, forse è meglio) di rientrare sulla giusta strada - potrebbe riconfermare la stessa condotta scorretta, e questo noi lo temiamo. Anche dal vaglio della Camera il testo del decreto-legge esce quindi sostanzialmente immutato. Al termine del suo *iter*, il decreto-legge evidenzierà una sua paradossale contraddizione, quella di essere nient'altro che un condono: anche se voi dite che non è così, si tratta di un condono a favore delle aziende che, indifferenti alle regole imposte dall'Unione europea e dalla legge n. 119 del 2003, hanno agito all'insegna dell'arbitrarietà.

In 40.000 hanno contenuto la produzione secondo le regole, hanno speso centinaia di milioni di euro per acquistare le quote latte ed ora saranno invece premiati coloro che si sono comportati in modo scorretto, soprattutto nei riguardi di chi si è indebitato per mettersi in regola, di chi ha fatto sforzi veri, di chi ha affittato le quote, cercando anche forme diverse, ma comunque onerose, per regolarizzarsi. Se le modifiche apportate al Senato non sono state sufficienti a farci cambiare opinione, quelle non apportate alla Camera hanno rafforzato la nostra idea: si è mantenuta l'impostazione del decreto-legge, e pertanto, così com'è, il testo non tranquillizza i cosiddetti regolari; e figuriamoci se può tranquillizzare noi! Non veniteci a dire che abbiamo dato retta alle associazioni di categoria: vorrei che nessuno dimenticasse che le associazioni riportano la voce dei propri associati e che quindi sono degne di considerazione. Non diteci, quindi, che il decreto-legge risolverà la questione. Abbiamo visto le associazioni in piazza qui e a Montecitorio,

il Parlamento. Così facendo, signor Ministro, state elaborando un decreto-legge per pochi, quando la maggior parte delle imprese agricole sono a rischio. Occorrono interventi tempestivi a sostegno degli agricoltori, ma si rileva una modesta attenzione da parte del Governo verso questo settore primario dell'economia italiana, che risente oltretutto della forte competitività a livello internazionale. Questo, Ministro, lei lo sa, ma avete preferito garantire molte opportunità a pochi eletti, anziché fondamentali necessità a tutti gli allevatori che in questo Paese

*(PD)*. Signor Presidente, cercherò di essere molto sintetica. Colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, in questi ultimi giorni e nelle difficili ore che vive l'Italia, stiamo avendo, proprio dal Paese e nel suo dramma, segnali positivi con la straordinaria solidarietà di ogni cittadino e cittadina verso i colpiti dal dramma del terremoto e con la competenza e la velocità dei soccorsi. A parte ciò, da ogni forza politica, specialmente dai partiti dell'opposizione, c'è stato grande senso di responsabilità e la consapevolezza che di fronte alle tragedie, al lutto e al dolore non c'è una parte, non c'è un colore, ma il dovere di tutti di concorrere al ritorno alla normalità. Anche il Presidente del Senato, il senatore Schifani, con parole giuste ed adeguate oggi lo ha riconosciuto nell'intervista rilasciata al «Corriere della Sera». Dunque, di fronte ai gravi problemi dell'Italia e alle sue sofferenze deve esserci un concorso di aiuti e di sostegni. Tuttavia, oggi - lasciatemelo dire - davanti all'ennesimo decreto-legge del Governo e all'ennesima richiesta di fiducia, viviamo una stridente contraddizione con il clima esterno e con quell'appello che ci viene da così alta carica. Qui c'è un atto unilaterale che non può essere modificato né migliorato. È stato sottolineato da molti come questa sia una ripetuta mortificazione del Parlamento, delle sue prerogative e della sua stessa valenza. Le assicuro, signor rappresentante dover vivere una simile condizione, vedersi sottratta la possibilità di dare un pur minimo contributo, di avanzare una piccola proposta per migliorare la condizione del Paese. Non c'è la possibilità di avere un dibattito vero e proprio, aperto, per trovare le soluzioni più adeguate.

e alla quale molto spesso ci si è richiamati in questi tempi, in queste settimane, cioè quella del «si salvi chi può» e con un metodo sbagliato: puntare sull'offerta invece di leggere, ascoltare o interpretare la domanda che viene dal Paese. Siamo di fronte ad un Esecutivo che non dà risposte alle domande e propone risposte dove non ci sono né domande né necessità.

Le domande vere sono quelle che provengono da un Paese in difficoltà, nel quale da un anno si è abbassata la produzione industriale, hanno chiuso molte aziende, è aumentato il ricorso alla cassa integrazione, è cresciuta la disoccupazione ed interi settori sono entrati in grave difficoltà. L'insieme di questi fattori ha avuto ripercussioni negative sulla distribuzione dei redditi e sulle buste paga, con le famiglie che si sono viste aggiungere ai problemi di sempre quelli derivanti dalla cassa integrazione guadagni, dalla perdita dei posti di lavoro e dal diminuire delle possibilità occupazionali per i loro figli, quei giovani ai quali non basta dire di darsi da fare e di non stare con le mani in mano. A quei giovani non basta fare questi appelli! Le persone che vivono in una condizione di povertà - che non sono poche nel nostro Paese - si sono ulteriormente impoverite. Qual è dunque il progetto sociale che il Governo ha in mente, quello al quale il Presidente del Consiglio pensa quando dice che non lasceremo solo nessuno in questa crisi? A queste domande, a queste famiglie, a questi disoccupati bisogna dare risposte adeguate e concrete

poi, aiuta le aziende automobilistiche. Ma che effetti hanno avuto gli altri provvedimenti in questo senso? Perché il Governo non viene a dirci quali sono i risultati? Dobbiamo apprendere le notizie dai giornali senza avere un'analisi, un

Abbiamo fatto - lo dico davvero in pochi secondi - due proposte. La prima sulla riproposizione del credito d'imposta, che serve, che è un aiuto virtuoso, che è strumento per allocare correttamente le risorse e per premiare le imprese in modo trasparente.

stornati e utilizzati per altro. Anche questa volta non s'è voluto dare questo segnale positivo.

alla fiducia ci si sia espressi nel complesso e lo si sia adeguatamente approfondito. Questa è la ragione per cui tratterò esclusivamente di un punto particolarmente significativo di questo decreto, vale a dire l'articolo 7-*octies*, che riguarda il rimborso dei titoli azionari Alitalia. Parlo specificatamente di questo problema perché la questione riguarda non poche persone, ma 40.000 obbligazionisti italiani a cui si aggiunge un congruo numero di azionisti. In buona sostanza, parliamo di una questione che riguarda piccoli risparmiatori che complessivamente hanno investito quasi 600 milioni di euro in questa partita.

gli obbligazionisti debbano oggi scegliere al buio: in sostanza, hanno novanta giorni di tempo per scegliere se aderire o meno a questa offerta pubblica di scambio e mi chiedo: perché adesso, considerato che la trattazione delle domande di ammissione allo stato passivo è fissata per il 21 ottobre prossimo? Sarà quella la data in cui sapremo effettivamente quale è la quota di recupero e che cosa effettivamente può essere a disposizione dei creditori. Perché non posticipare di qualche mese la soluzione del problema, visto che la materiale disponibilità delle risorse agli obbligazionisti che aderiscono comunque andrà materialmente dopo quella data?

Alitalia avrà risorse da portare casa. Aquesto punto chiediamo che quelle risorse siano destinate agli obbligazionisti a cui oggi viene sostanzialmente proposto uno scambio tombale, con la perdita di ogni diritto. E la consegna della totalità dei titoli conferma quanto dico. Infatti, poiché è previsto un rimborso non superiore a 100.000 euro per ogni obbligazionista, c'è la clausola, peraltro curiosa, che prevede che l'obbligazionista che si trova in mano il doppio

un argomento che ho tentato più volte, so anche che il sottosegretario Giorgetti lo conosce perfettamente e so che però, purtroppo, i tecnici del Ministero dell'economia continuano a ragionare in termini assolutamente strani rispetto a questa necessità.

nel resto d'Italia succede il contrario. Ma che Paese è questo? È un Paese dove tutti i cittadini sono di serie A, o ci sono cittadini di serie A, di serie B e serie C? È giusto che la collettività paghi per i rifiuti dei cittadini di Palermo, in una situazione economica di questo tipo? E poi diciamo al lavoratore che ha perso il lavoro e che ha pagato le tasse fino a ieri, che era dipendente di una piccola impresa e quindi non ha diritto alla cassa integrazione, che per lui non c'è alcuna risorsa.

Esiste un comma che prevede che si sblocchi il Patto di stabilità con una somma veramente ridicola, che ha un limite di 150 milioni di euro. In questo modo non si fa altro che prendere in giro gli italiani le amministrazioni locali, che avevano applaudito a quella nostra iniziativa *bipartisan*, perché tutte le forze politiche si sono vantate di quel provvedimento, mentre concretamente nonsiamo riusciti a tirar fuori "un ragno dal buco". il nostro Paese possa venir fuori da questa situazione e possa venirne fuori più forte, perché nei momenti di difficoltà gli italiani hanno sempre dimostrato di riuscire a vincere le sfide.

questa legislatura al Senato. Basti pensare che Prodi, nello stesso periodo, ne aveva collezionate ben otto. Tanto meno ci scandalizza l'utilizzo dello strumento del decreto-legge, perché solo un marziano potrebbe non riconoscere la necessità e l'urgenza che devono caratterizzare l'azione del Governo e del Parlamento, soprattutto in una fase così delicata sotto il profilo sociale e finanziario. Il presidente Berlusconi, qualche giorno fa, si è nuovamente soffermato su un importante concetto: il Governo non lascerà indietro nessuno. E non è stato un esercizio di ottimismo, che pure è determinante coltivare, bensì la plastica rappresentazione dell'obiettivo che questo Governo e la sua maggioranza si sono posti, di fronte ad una crisi che è di portata mondiale e che non ha alcun precedente. Riteniamo corretto che l'ottimismo gratuito non contagi le previsioni e le stime scientifiche modulate da istituzioni internazionali; ma paradossalmente riscontriamo l'inesistenza di una *exit strategy* (a livello globale, ovviamente), della quale dovrebbero farsi promotrici proprio istituzioni come l'OCSE, la Commissione europea o il Fondo monetario, che invece dispensano segnali di pessimismo cronico ma non offrono originali soluzioni, né tanto meno indicano qualche terapia. L'emergenza è ora. Il bollettino dei danni è assai noto. Occorre quel sano pragmatismo attuato in Italia dal centrodestra e condividiamo pienamente il pensiero del *Premier*, quando dice che dobbiamo difendere in primo luogo i disoccupati e poi ci occuperemo dei vincoli imposti da Bruxelles. A chiunque dei venti milioni di disoccupati che probabilmente si materializzeranno quest'anno nel mondo interessano poco le fredde percentuali o le rigide statistiche elaborate dalle citate istituzioni internazionali. Ai disoccupati, ai cassintegrati, alle famiglie e alle imprese interessano molto di più provvedimenti come quello attualmente in discussione, che non ha certamente la presunzione di essere la panacea per tutti i mali, ma che è senza dubbio un importante tassello nel mosaico strategico anticrisi varato dal Governo. Il *bonus* previdenziale per chi assume i lavoratori posti in cassa integrazione o che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi rappresenta un'azione di sostegno certamente

Accelerare i tempi per la concessione della cassa integrazione attraverso l'INPS, ad esempio, è un'altra risposta positiva alla richiesta d'aiuto che proviene dal mondo del lavoro e dai sindacati.

quindi l'incentivo di antica memoria al quale eravamo abituati. Questa politica di aiuto al settore dell'auto, che un tempo significava riaffermare quella che era diventata quasi una dottrina della socializzazione delle perdite e della privatizzazione degli utili, ma solo in casa FIAT, oggi ci consente di manifestare anche un moderato orgoglio per l'inusuale ruolo che l'industria automobilistica italiana si trova a svolgere sullo scenario internazionale.

Pensiamo che intervenire positivamente anche sulle detrazioni fiscali per l'acquisto di elettrodomestici e di mobili sia la strada migliore per restituire fiducia nel futuro a tutti gli italiani che abbiano deciso di ristrutturare un immobile, cioè di mettersi in gioco anche economicamente, e alle imprese che producono e commercializzano tali prodotti. Questo è il momento di intervenire per ridare speranza alle famiglie, per sostenere la domanda e le imprese di qualsiasi dimensione, per aiutare le banche sane, il cui ruolo è delicato e importante soprattutto in questa fase temporale. E quando dico che questo provvedimento è un'ulteriore tessera di un complesso mosaico di interventi a favore dell'economia, intendo implicitamente ricordare - mi fa piacere che in Aula sia presente il sottosegretario Alberto Giorgetti - quello che è accaduto nel recente passato e che sta accadendo sulla scorta di una legge finanziaria rigorosa, a volte impietosa, forse anche impopolare, ma estremamente attenta alla valorizzazione e alla tutela del risparmio, alla riorganizzazione del sistema Paese. Cito, ad esempio, il sostegno alla diffusione della banda larga, al trasporto su ferro, all'apertura dei cantieri indispensabili per le grandi opere, alle semplificazioni burocratiche, al riordino degli incentivi in materia energetica non più sui programmi, ma questa volta sui progetti; per non parlare della detassazione degli straordinari o della riduzione del carico fiscale sulla prima casa. poste in essere tentando ovviamente di mantenere invariato il debito pubblico che abbiamo ereditato dai sollazzi della prima Repubblica. Il testo in esame contempla un intervento a favore della filiera del tessile relativo all'istituzione di un Fondo di garanzia di 10 milioni di euro, anche in questo caso legato alla questione ambientale, cioè allo smaltimento dei rifiuti ed alla depurazione delle acque. È il primo intervento di quella che si prospetta come una lunga serie a favore del tessile. Un segnale importante che accompagna questo decreto è l'avvenuta costituzione del tavolo moda, inteso come laboratorio per la discussione dei problemi che stanno attanagliando il mondo del tessile e dell'abbigliamento e l'elaborazione di successive e conseguenti proposte. Stiamo lavorando per il credito di imposta per la realizzazione dei campionari e delle collezioni, o per i progetti innovativi finanziati col Fondo per l'innovazione tecnologica o le misure per promuovere prodotti certificati in termini di eco-compatibilità e sicurezza. Il tessile abbigliamento in Italia occupa direttamente - poi vi è l'indotto - più di 500.000 addetti ed ha un fatturato che passa abbondantemente i 54 miliardi di euro e dalla sua ripresa dipendono i destini non solo dell'indotto poco fa citato, ma anche degli operatori del commercio. Occorre fare di più intervenendo ad esempio in materia di lotta alla contraffazione, ma so contraffatti sequestrati nel 2008 sono il doppio di quelli sequestrati nel 2007; quindi, il Governo è presente anche in questa materia e occorre fare di più anche sulla tutela del lavoro femminile. Il settore tessile non ha l'abitudine di chiedere aiuti ed in passato è stato anche penalizzato dalle scelte dell'Unione europea e da una concorrenza sleale del Sud-Est asiatico. Comunque, il provvedimento in discussione è attento ed ha recepito anche proposte avanzate dai parlamentari: da lombardo non posso dimenticare che questo testo recepisce le indicazioni che ho elaborato con alcuni colleghi del PdL in relazione alla salvaguardia del trasporto pubblico lacuale, sul lago di Como, sul Garda. Lo sa molto bene anche l'onorevole Giorgetti, veronese, che ha seguito con noi questo tipo di provvedimento. La finanziaria aveva messo a repentaglio parecchi posti di lavoro e soprattutto l'economia del turismo, che in Lombardia si fonda anche sulle bellezze artistiche e naturali dei laghi prealpini. Oltretutto il trasporto lacuale è anche una valida alternativa al tradizionale trasporto su gomma. Ebbene, il nostro ringraziamento va - come dicevo - all'onorevole Giorgetti, ma particolarmente al ministro Matteoli, ai dirigenti del suo Ministero ed anche all'Ente governativo gestione dei laghi perché sono stati ottimisti e propositivi. Grazie a questo tempestivo intervento non ci sono stati ridimensionamenti del personale e soprattutto delle corse dei battelli, con buona pace anche dell'industria del turismo, pesantemente in crisi anche in Lombardia. La situazione è critica, ma anche in virtù di provvedimenti come quello in esame il mondo dell'impresa risulta oggi assai meno pessimista rispetto a soli tre mesi fa. La maturità e la responsabilità di un sistema si misurano anche attraverso la serenità, la puntualità e la competenza con cui si lavora tutti insieme, se possibile, per sconfiggere il più rapidamente possibile gli effetti di una crisi mondiale senza precedenti.

il prossimo 28 aprile l'Aula del Senato inizierà a discutere, in terza lettura, il disegno di legge delega sul federalismo fiscale. Si tratta di un appuntamento importante e da tempo atteso, poiché finalmente si dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione che prevede l'autonomia finanziaria per le Regioni e gli enti locali. Il Gruppo del PD ha fortemente contribuito a definire il testo approvato dalla Camera, che ora è molto diverso da quello inizialmente proposto dal Governo e prevede molte delle norme contenute nel nostro disegno di legge. Ma ciò che colpisce in modo clamoroso è la distanza siderale tra la volontà annunciata, quella cioè di realizzare il federalismo fiscale, e la politica rigidamente centralistica del Governo, che attua nei confronti delle autonomie locali un atteggiamento di totale chiusura alle loro istanze come raramente si era visto anche in passato. Non basta invocare i vincoli di finanza pubblica, che conosciamo bene e che noi per primi proponiamo di assumere responsabilmente. La verità è che l'approccio del Governo alla crisi economica e al tema stesso del Patto di stabilità interno sono completamente sbagliati. Ormai questa è una consapevolezza che ci accomuna ad alcune forze della maggioranza, a cui ci appelliamo perché si uniscano a noi nel pretendere un cambiamento radicale dell'atteggiamento del Ministero dell'economia. Il Governo si illude di governare centralmente la finanza locale, negando ai Comuni, compresi quelli virtuosi, persino la possibilità di effettuare i pagamenti per le opere già appaltate. La realtà dimostra che molti enti locali saranno costretti, dalla miopia di questa assurda pretesa del Governo, a non rispettare i limiti del Patto di stabilità interno, con conseguenze ancor più negative per i conti pubblici. Anche le associazioni d'impresa e i sindacati, allarmati per una crisi economica gravissima, hanno chiesto con forza di allentare i vincoli sugli investimenti dei Comuni. È evidente che le grandi opere, molto lontane nel tempo, possono ben poco. Mentre per dare respiro alle imprese e ai lavoratori occorre un piano di medie e piccole opere, attivate dai Comuni, che siano immediatamente cantierabili. Anche la messa in sicurezza degli edifici pubblici, che sarebbe comunque stata necessaria ma la cui indilazionabilità è richiamata dal gravissimo terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila, può essere effettuata solo dando la possibilità a Comuni e Province di investire. La schizofrenia del Governo e della maggioranza è arrivata fino ad approvare, il 17 marzo scorso alla Camera, la mozione Franceschini sull'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per gli investimenti dei Comuni, che poi è stata puntualmente disattesa con l'articolo 7-*quater* del decreto-legge che stiamo ora discutendo. Nella mozione approvata alla Camera vi sono, in particolare, due impegni che risultano del tutto disattesi. riferisco all'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009 e all'esclusione dai saldi finanziari dei pagamenti effettuati con i residui passivi per spese di investimento nei limiti della disponibilità di cassa. Il decreto-legge subordina questa possibilità all'autorizzazione della Regione di appartenenza, la quale deve a sua volta rideterminare il proprio obiettivo programmatico ed il vincolo risulta talmente forte da rendere estremamente limitati ed incerti gli importi effettivamente disponibili a tale scopo. L'assurdità di questa situazione è che non si chiede di trasferire agli enti locali nuove risorse, ma di poter utilizzare una parte di quelle che essi hanno già. Gli avanzi di amministrazione dei Comuni ammontano a 3,2 miliardi di euro ed i residui passivi a circa 15 miliardi di euro, che sono immediatamente spendibili. Questa mattina il nostro Gruppo aveva dichiarato la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti, tranne quattro relativi al Patto di stabilità interno per gli enti locali. Avevamo proposto di sbloccare gli investimenti per 1,5 miliardi di euro, prevedendo la relativa copertura finanziaria. Il Governo ha posto ugualmente la questione di fiducia, che a questo punto risulta del tutto superflua, evidentemente perché non ha fiducia nella sua maggioranza e teme che una parte di essa possa sostenere i nostri emendamenti; ma sulle mozioni e gli ordini del giorno che presenteremo sul federalismo fiscale il Governo non potrà mettere la fiducia. Il Consiglio nazionale dell'ANCI, signor Sottosegretario, il 26 marzo scorso, ha approvato un documento nel quale si dice che l'attuale situazione è assolutamente straordinaria e, in ragione di ciò, si ritiene condivisibile il comportamento di quei Comuni che si troveranno a non poter rispettare il Patto di stabilità interno per il 2009. Noi insisteremo nel proporre ciò che contenevano gli emendamenti che oggi ci avete impedito di mettere in votazione, ma proporremo anche, se si continuerà così, di effettuare una sospensione selettiva delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno dovuto a spese di investimento da parte degli enti locali, previa una verifica, da fare entro giugno, dell'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica. Crediamo infatti che ci sia un interesse generale del Paese e della sua economia che va salvaguardato ad ogni costo, anche contro l'ostinato comportamento del Governo, che lo continua pervicacemente a negare.

due semplici considerazioni di due grandi premi Nobel per l'economia. La prima è di Amartya Sen, che ricordo con particolare rimpianto in un'Aula del Senato vuota. Amartya Sen, che si è trovato più volte di fronte a crisi

è utile alla politica economica perché consente di correggere gli errori che la politica economica può compiere. È una banalità; la democrazia è il confronto delle posizioni, delle idee, è il reciproco rispetto, è l'ascolto reciproco,

abbiamo votato un Documento di programmazione economico-finanziaria e la relativa finanziaria in poche ore, in un Parlamento che aveva bisogno di fare presto, perché si prevedeva una grande crisi globale della domanda. Forse non era vero, o forse era semplicemente una percezione particolare (una delle tante che coinvolgono spesso i pensieri molto contraddittori del nostro Ministro dell'economia)

non era forse l'impostazione del nostro Governo dal 2001 al 2006, quando si derubricava il reato di falso in bilancio delle aziende? Non era forse la nostra impostazione quando si incentivavano gli italiani a fare il secondo mutuo sulla casa per consumare di più, perché questo era necessario per mantenere salda e stabile la domanda? Non avevamo - lo direi da economista - una particolare affezione per la domanda in quei momenti nei quali essa non si sosteneva con una capacità di produzione crescente del PIL, ma si sarebbe sostenuta soltanto con strumentazioni finanziarie? Ebbene, ciò che sta accadendo non era così imprevedibile; del resto, ce lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti. Era imprevedibile che quello che stava accadendo dovesse mettere in discussione i presupposti generali della politica economica

- c'è una recessione o un'economia della depressione, l'unica modalità per affrontare situazioni di questo genere è immettere denaro nei mercati e fare in modo che i mercati, cioè la domanda, riprendano fiducia verso l'offerta, consentendo che si rimetta in moto un circuito positivo. Ci è voluto qualche mese per capirlo.

Ma quanti hanno notato la contraddittorietà di questo con altri discorsi che ha fatto

Non è questo che sosteneva il Partito Democratico qualche settimana fa, quando ha detto che si doveva mettere un punto di prodotto interno lordo al servizio di

quando non si usa la democrazia, non si correggono gli errori, gravi, che si stanno compiendo. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio esprimere il mio forte disappunto per il metodo adottato dal Governo. Siamo chiamati ad esprimerci sull'ennesimo decreto-legge e, come se ciò non bastasse, sull'ennesima richiesta di fiducia posta su un provvedimento importante per le sorti dell'economia di questo Paese, in quanto volto a sostenere i settori industriali in crisi. Con l'imposizione della questione di fiducia il Governo ha nuovamente soffocato il dibattito parlamentare e reso inutili tutti i nostri sforzi e le nostre proposte emendative per migliorare il testo. Ciò che mi trova assolutamente contrario è che in questo decreto siano confluite le nuove norme sulle cosiddette quote latte. Entrando nel merito del provvedimento, saluto con favore le misure in esso contenute volte al sostegno di alcuni di quei settori industriali fortemente colpiti dalla crisi. Reputo dunque positive le norme volte ad aumentare la domanda, attualmente fortemente compromessa. A tale riguardo penso ai *bonus* per la rottamazione di auto, moto ed elettrodomestici; assai positivo anche il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che potranno contare anche sul sostegno della Cassa depositi e prestiti. Saluto poi con favore il pacchetto per i precari, le norme contro la contro la speculazione in Borsa, nonché le misure sulle pensioni per i lavoratori esposti all'amianto. tutto ciò è troppo poco per rilanciare effettivamente l'economia e per sostenere effettivamente le

devo evidenziare la totale mancanza di misure a sostegno del settore turistico, anch'esso fortemente colpito da questa crisi e nei confronti del quale la politica continua a non dare risposte concrete. Mi preme, a tale riguardo, ricordare che in Italia il settore del turismo ha da tempo perso il suo primato storico nel mondo. Diversamente da altri settori economici, gli operatori del turismo non possono risparmiare delocalizzando; mi preme sottolinearlo, perché questo settore garantisce migliaia di posti di lavoro che vengono messi a repentaglio da questa crisi e che meriterebbero maggior attenzione e sostegno da parte del Governo. Un segnale di sostegno da parte del Parlamento fortunatamente c'è. Alludo al disegno di legge n. 1301 relativo a nuove disposizioni in materia di turismo, attualmente all'esame della Commissione di istituzione di un Ministero delle politiche turistiche, riconosce il significato strategico delle politiche di *marketing* integrate. Mi auguro che questo disegno di legge, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori, possa essere discusso in modo approfondito ed approvato dal Senato in tempi rapidi, al fine di dare un contributo al settore del turismo e quindi al rilancio economico complessivo del Paese. Un altro problema che mi preme segnalare è l'eccessiva severità dei controlli in alcune Regioni, soprattutto del Nord, che rischia fortemente di alterare ed incrinare il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini in generale e tra fisco ed imprese in particolare, fatto che in altre Regioni ciò non accade. La necessità di fare emergere il lavoro sommerso, di combattere l'evasione fiscale e di garantire la sicurezza sul posto di lavoro è fuori discussione. Tuttavia, ciò può e deve avvenire senza che le piccole medie imprese vengano messe sotto torchio. In un momento così delicato serve un fisco più amichevole, che accompagni le aziende con consulenze al fine di creare una cultura contributiva corretta. Occorre, insomma, un nuovo metodo accompagnato

i disonesti penalizzando chi in questi anni ha rispettato le regole anche a costo di indebitarsi. Ciò che mi ha fortemente deluso è che alla Camera, in sede di conversione, sia stata esclusa dal maxiemendamento del Governo la norma sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Lo scorso lunedì questa norma è stata trasformata alla Camera, in Commissione agricoltura, in un disegno di legge; al fine di ottenere una rapida approvazione, la Commissione ha avviato la procedura per il trasferimento in sede legislativa. Mi auguro fortemente che il Governo e le Commissioni diano parere favorevole per risolvere una volta per tutte un problema che si trascina ormai da mesi.

voglio esprimere, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, la mia solidarietà ai miei corregionali, colpiti dal gravissimo terremoto di questi giorni, e il mio cordoglio per le tante vittime. Auspico che in una situazione come questa tutti noi ci impegniamo al massimo, lasciando per un attimo da parte le polemiche e i distinguo politici, per fare in modo che alle popolazioni colpite arrivi in breve tempo necessario sostegno materiale e morale affinché, passati i giorni del dolore e del lutto, l'Abruzzo tutto possa rialzarsi e ricostruire quello che la forza della natura ma anche, lasciatemelo dire, la superficialità dell'uomo che in nome del profitto non ha seguito le dovute norme, hanno raso purtroppo al suolo. Nonostante la crisi in atto, è necessario trovare subito le risorse e agire in fretta affinché non capiti, come in altre regioni colpite da catastrofi analoghe, che una volta scomparsa la notizia dai giornali ci si dimentichi dei sopravvissuti. Tornando al provvedimento in discussione, devo purtroppo stigmatizzare le modalità d'intervento del Governo rispetto a questa crisi. Siamo di fronte al trentacinquesimo decreto varato da questo Governo e alla quindicesima richiesta di fiducia in 11 mesi, sommando quelle della Camera e del Senato. Una decretazione utilizzata spesso senza che ci siano la necessità e l'urgenza previste per questo tipo di provvedimento. Ancora una volta, in un momento così delicato per il Paese, si impedisce al Parlamento di dare il proprio contributo tramite un'ampia discussione, ed eventuali modifiche o integrazioni, a scelte importanti per la nostra economia. Inoltre, il maxiemendamento introdotto alla Camera dei deputati lo ha reso un decreto *omnibus*, dal contenuto fortemente disomogeneo che va dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del Fondo di garanzia per le imprese, passando per i micro rimborsi per i risparmiatori Alitalia alle quote latte e agli ammortizzatori sociali. Un *pot-pourri* che va a modificare provvedimenti appena approvati e che ripropone parte di decreti scaduti come quello sulle quote latte che premia - l'ha già detto stamattina un mio collega - quei pochi allevatori che non ha hanno rispettato la legge e penalizza i tanti onesti. L'atteggiamento di questa maggioranza su molti argomenti si dimostra fortemente contraddittorio. Voglio ricordare che solo la settimana scorsa questa Assemblea ha bocciato due mozioni: quella del mio Gruppo, l'Italia dei Valori, e quella del PD che si richiamavano agli impegni di Kyoto per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici ha invece approvato una mozione che di fatto nega ciò che è stato riconosciuto dagli scienziati di indiscutibile fama dell'IPCC, la principale organizzazione internazionale in tema di cambiamenti climatici, che individuano nelle attività umane una delle cause principali del riscaldamento globale. Per contro, troviamo in questo decreto delle norme che potremmo definire ecologiche e che si richiamano a quelle varate dal Governo Prodi, come gli incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti con altri meno inquinanti e l'incremento dei vigenti incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici e per l'installazione di impianti a metano o a GPL. Peccato però che, all'articolo 5-*bis* dello stesso decreto, ci troviamo di fronte alla schizofrenia ambientale di questo Governo. Con questa norma, infatti, si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche ad olio combustibile in nuove strutture a carbone, non solo per i nuovi progetti ma anche per i procedimenti già in corso come, ad esempio, la centrale di Porto Tolle all'interno del Parco naturale del Delta del Po. È purtroppo risaputo che il carbone non è un combustibile amico dell'ambiente, a causa dell'acido solforico che forma con i fumi emessi dalle fornaci, per non parlare del fatto che tale norma prevede una deroga alle vigenti leggi regionali in materia, con buona pace dell'appena approvato federalismo. L'unico aspetto certo è che mentre in tutto il mondo il contrasto ai cambiamenti climatici e le politiche ambientali stanno diventando una delle voci maggiori dell'economia (basti pensare che in Europa sono già oltre 4 milioni i posti di lavoro legati alle politiche ambientali, alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alle bonifiche ambientali, si prevede che entro il 2020 diventeranno 8 milioni), in Italia si negano i cambiamenti climatici e invece di legare le ragioni del lavoro e dell'economia a quelle dell'ambiente, si fa in modo che su questi temi diventi il fanalino di coda non solo in Europa ma nel mondo. Anche per quanto riguarda il lavoro, gli interventi del Governo non sono assolutamente sufficienti. Sembra che il Governo si sia accorto della gravità della crisi e dei suoi tragici effetti sui lavoratori solo dopo il recente Vertice dei Ministri del lavoro del Purtroppo, i dati dell'OCSE parlano chiaro. Infatti, se i dati per il 2009 non sono confortanti, le previsioni per il 2010 sono veramente preoccupanti: ci sarà un ulteriore calo del PIL, un ulteriore calo della domanda interna e un aumento del tasso di disoccupazione, che raggiungerà il 10,7 I dati resi noti ieri dall'INPS li abbiamo letti tutti e sono davvero impressionanti: solo nel primo trimestre del 2009 la richiesta di indennità di disoccupazione è aumentata del 45,9 750.000 domande contro le 520.000 del 2008. Allo stesso modo, è aumentato il ricorso delle imprese alla cassa integrazione. La cassa ordinaria, infatti, nel solo mese di marzo ha avuto un vero e proprio *boom*, con un aumento del 925 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008 e - pensate - del 589 per cento nel primo trimestre sempre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Interi settori nevralgici della nostra economia, come la metallurgia e l'edilizia, stanno ricorrendo alla cassa integrazione in modo esponenziale. Non è pensabile affrontare una crisi di questa portata senza prevedere interventi strutturali in materia di lavoro, a partire - continuiamo a ripeterlo - da una riforma organica degli ammortizzatori sociali: fino ad oggi ci sono stati solo interventi frammentari. Con questo provvedimento sugli ammortizzatori sociali in senso stretto si va verso un piccolo miglioramento della cassa integrazione in deroga, ma siamo lontanissimi dalla richiesta che si introduca un ammortizzatore di tipo universale. inoltre vero che viene salvaguardata l'autonomia contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma avremmo voluto che il Governo avesse previsto, per gli accordi sulle crisi da affrontare con la cassa integrazione in deroga, degli incentivi per mantenere in attività la gran parte dei lavoratori interessati, evitando l'utilizzo della cassa integrazione a zero ore e promuovendo i contratti di solidarietà, come abbiamo sottolineato nella nostra mozione. Anche per i co.co.pro. c'è un miglioramento, ma si mantengono le diversità strutturali di trattamento rispetto agli altri contratti; la loro natura di contratti di lavoro dipendente, dissimulati sotto la veste del lavoro atipico, purtroppo rimane tutta. Sempre all'articolo 7-*ter*, al comma 7, è previsto un *bonus* previdenziale a favore delle imprese non in crisi che assumano lavoratori sospesi o estromessi dal mercato del lavoro per crisi aziendale. L'interpretazione più pessimistica di questo comma porterebbe alla conclusione che tale beneficio spetterebbe solo alle aziende *ex* articolo 1 della legge n. 223 del 1991, *ergo* quelle con più di 15 dipendenti. Se così fosse, anche in considerazione del fatto che il sistema italiano delle imprese è costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, si tratterebbe di una grande limitazione alla ricollocazione di manodopera, soprattutto in una fase storica come questa. Siamo quindi davanti ad interventi frammentati e marginali che partono da una visione del Paese limitata, che non danno risposta a chi non ha abitazioni da ristrutturare o auto da acquistare ma che vorrebbe semplicemente lavorare e poter contare alla fine di ogni mese su un salario che gli permetta di vivere dignitosamente o sul sostegno economico nel momento o sul sostegno economico nel momento in cui, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dal tipo di contratto stipulato, il lavoro purtroppo non lo ha più. *(Applausi

prassi, fu fatta una ricognizione, una valutazione della produzione lattiera, una specie di censimento produttivo, ignorando forse volutamente, forse anche per errore, una miriade di piccole e piccolissime imprese che producevano latte a livello artigianale.

Non so se questi agricoltori allora furono volutamente ignorati dal Governo Craxi, che aveva maggiore interesse a sostenere le produzioni industriali a discapito di quelle agricole. A noi quel che interessa oggi è che purtroppo

che, senza alcun tipo di certificazione, entra illegalmente nel nostro paese. Credo che da parte di tutti vada riconosciuto il gran lavoro dei ragazzi della Guardia di finanza che svolgono ottimamente il loro compito.

Fu allora che iniziò questa triste storia. Fu allora che iniziò la genesi delle quote latte. Oggi stiamo cercando di sistemare le cose, non con le solite parole e la solita demagogia politica, politica, ma con i fatti concreti, con la sostanza e la concretezza del lavoro e dei risultati ottenuti dal ministro Zaia a Bruxelles. Con questo decreto - lo abbiamo detto diverse volte - riusciamo a distribuire 640.000 tonnellate di quote latte, pari al 6 per cento della produzione. Una notevole quantità, ottenuta grazie al lavoro del Ministro che finalmente ha spostato l'attenzione della Comunità europea verso la nostra agricoltura. Un provvedimento, questo, che è una risposta con i fatti a chi critica, sempre e costantemente, speculando sulle difficoltà di tante aziende agricole che rischiano di chiudere la loro attività. Alla Lega non interessa il percorso istituzionale, non interessa se è giusto o corretto parlare di quote latte insieme agli incentivi per la rottamazione, non interessa se questo viene fatto con un decreto piuttosto che con un disegno di legge.

a noi interessano in particolare le zone di montagna; interessa il Fondo di garanzia per chi ha acquistato le quote in passato; a noi interessano le oltre 8.400 aziende, che purtroppo rischiano concretamente di chiudere. Oggi, invece, queste aziende possono salvarsi da un sicuro fallimento dilazionando il loro debito. Sicuramente manca il Fondo di solidarietà, lo abbiamo detto un po' tutti, ma anche per quanto riguarda quest'ultimo nei prossimi giorni credo che troveremo una soluzione. In Commissione agricoltura abbiamo già trovato l'accordo. Il futuro passa comunque attraverso una revisione verso l'alto dei prezzi dei prodotti agricoli. Credo che di fondamentale importanza sia il vertice dei Ministri dell'agricoltura che si terrà tra una decina di giorni, finalmente in Italia,

affermando che questa è la politica del fare e per questo motivo la Lega Nord voterà a favore Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, il dibattito di questa giornata è segnato - non poteva essere diversamente - dalla mestizia per i tragici eventi occorsi in Abruzzo. se riflettiamo e pensiamo a questa giornata, c'è anche uno svuotamento, uno svilimento del ruolo di quest'Aula. Se non vado errato, ci troviamo per la sesta volta a discutere di un provvedimento di misure urgenti in campo economico, senza avere avuto alcuna possibilità di interagire nel merito sui contenuti di quel provvedimento.

Non è il Parlamento che non funziona (ci aspettiamo una delle solite intemerate): ieri, ad esempio, la 6a e la 10a Commissione riunite, pur nel breve spazio consentito per poter discutere su alcuni emendamenti, hanno svolto un confronto approfondito, con spunti interessanti. È il Governo, è la sua maggioranza che stanno sminuendo il ruolo di questo ramo del Parlamento, privandosi della possibilità di ottenere contributi, apporti, quello sforzo comune, solidale e coeso, necessario per fronteggiare una situazione di grande difficoltà, come quella che il nostro Paese sta attraversando. Venendo al merito, riteniamo condivisibili alcune misure contenute nel provvedimento, mentre altre sono del tutto da rigettare, ma denunciamo la loro inadeguatezza rispetto alla criticità dei problemi da affrontare. Non voglio farla lunga citando molti dati, ma gli ultimi riferimenti dell'ISTAT parlano da soli. A gennaio, gli ordinativi hanno fatto registrare un segno negativo del 31 per cento rispetto a 12 mesi prima.

orientativamente collocate tra il 2 e il 2,5 per cento di calo. È una situazione grave per la quale non bastano la fantasia e la volontà, ma sono necessari interventi decisivi, una visione organica e una strategia compiuta,

e un sostegno forte - com'è stato ripetuto in diversi interventi - sul piano degli investimenti, soprattutto al fine di porre in condizione gli unici soggetti che sono in grado di spendere e accantierare rapidamente (gli enti locali) di poter utilizzare le risorse che hanno a disposizione e che non possono essere messe in gioco per un rispetto formale del Patto di stabilità. Certo, viene spesso opposto

pubblici e di rigore finanziario ce ne intendiamo, visto che abbiamo contribuito in diverse circostanze al risanamento dei conti pubblici con significativi risultati, anche se non sempre ci sono stati riconosciuti. Il problema del debito è debito è importante, ma allo stesso tempo bisogna interrogarsi su come possano tenere i nostri conti senza fare politiche anticicliche di investimenti e di sostegno alla domanda e alle imprese. In altri termini, pensiamo che non si uscirà dalla crisi, riducendo al massimo i danni sociali e quelli relativi al patrimonio industriale del Paese, se non si fa attenzione a recuperare la capacità di tenuta del Paese, della sua solidità di insieme, del suo tessuto delle micro e medie imprese e della capacità lavorativa e professionale. Non sarà neanche possibile garantire la tenuta dei conti pubblici, e questo mi pare assolutamente evidente.

Ci vuole una strategia e non un profilo minimalista. Al contrario, si ha l'impressione che il Governo rincorra la crisi, cercando di tamponare le falle che di volta in volta la stessa crisi genera, invece che prevederne e governarne l'andamento. Nella crisi c'è anche un fattore tempo che è decisivo e c'è un altro aspetto molto importante che concerne il profilo degli interventi. Ad esempio, va

attiene alle ristrutturazioni edilizie e che è stato richiamato anche con riferimento alla questione del piano casa: dobbiamo affermare una serie di interventi che si muovano soprattutto nella logica dell'economicità, dell'ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente. Mi pare che questo profilo e questa intenzione non emergano. Così come non

che erano nella versione originaria della legge finanziaria 2006, poi modificate nel decreto-legge n. 112 che ora si modifica di nuovo, estendendo così la possibilità del consolidato e del concordato preventivo triennale anche alle imprese IRPEF e non solo IRES e anche ai tributi dovuti a livello locale; dall'altro, si estende tale agevolazione anche alle reti delle imprese e delle catene di fornitura, estensione che era stata adombrata, ma poi esclusa, nella stesura del decreto-legge n. 112. A fronte delle complessità e delle problematiche giuridiche, amministrative, economiche e contabili che emergeranno in fase di attuazione della norma, si prevede un tetto di soli 10 milioni di euro per il 2009 e di 50 milioni annui per gli anni successivi. E allora, delle due l'una: o il gioco non vale la candela o si vuole di fatto introdurre l'ennesima scappatoia fiscale per le imprese, posto che «in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio» (articolo 3, comma 2). Anche da questa impostazione e da queste misure, come da altre contenute nel decreto, emerge uno spaccato utile a delineare la strategia con cui il Governo si pone nei confronti del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale: ci sono misure lasche e il messaggio un po' l'occhio, è che «chi può, si arrangi». A dire il vero, questo provvedimento è anche un segnale di resipiscenza, perché si introducono, all'articolo 7, severe misure sanzionatorie nel caso le imprese, ad esempio nella compensazione dei crediti, si comportino in maniera non corretta. Certo, le grida vanno bene e i controlli anche, perché sono previsti controlli severi per accertare comportamenti eventualmente non lineari. Ma forse sarebbe stato meglio non cancellare le misure che un altro Governo e un altro Ministro, qualche tempo fa, avevano introdotto, ad esempio l'obbligo di comunicazione preventiva per poter compensare crediti di imposta superiori ai 10.000 euro, misura che aveva trovato la sua motivazione nella dinamica molto accentuata di quelle compensazioni, a fronte della consapevolezza che i più importanti

come quella della limitazione nell'uso dei contanti e degli assegni, la tracciabilità dei pagamenti, la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati, la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore. Ho richiamato questi temi perché,

è un dovere, non solo nei confronti dei cittadini che sono in condizioni di sofferenza nel loro potere di acquisto, ma anche nei confronti delle imprese, tra un'impresa che si comporta lealmente nei confronti del fisco ed una che si comporta in maniera impropria c'è una concorrenza sleale, che deprime l'impresa che normalmente è più sana e corretta, che andrebbe invece sostenuta. Mi auguro che arrivi finalmente il tempo in cui il Ministro dell'economia consegni al Parlamento quel rapporto, cui è tenuto da un obbligo di legge, circa i risultati del contrasto e della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, e che sia finalmente possibile in quest'Aula condurre una discussione seria, approfondita e di merito per prendere misure che vadano nella direzione di del Ministero e delle Agenzie competenti nel contrasto all'evasione e all'elusione, per restituire risorse che possono servire a ristorare i cittadini, abbassare la pressione fiscale e sostenere il sistema dell'economia e delle imprese nel nostro Paese.

un pensiero affettuoso ai fratelli della terra d'Abruzzo, per i quali questa sera siamo impegnati ad essere seri come si conviene e severi come necessario.

e siamo sul punto di approvarlo con un voto di fiducia necessitato, che il Governo avrebbe voluto evitare, ma al quale evidentemente ricorre nell'interesse superiore della Nazione e del processo legislativo, ad esso connaturale e necessario.

d'impresa. Il Governo è meritevole e di esso apprezziamo l'ansia e la frenesia con le quali, nei limiti del possibile, si appresta di volta in volta a soccorrere questo sistema produttivo e il nostro popolo nei suoi bisogni.

è poi la questione della scissione e della fusione. Il Governo ha eliminato, per questo periodo, il ricorso ai principi contabili internazionali; ha consentito che per questo esercizio non si debba necessariamente valutare i titoli al prezzo corrente, altrimenti avremmo dovuto mettere in liquidazione tutte le aziende d'Italia.

la rivalutazione sostitutiva dell'immobile, anche questa molto virtuosa e positiva, e la SACE, questa sorta di garanzia che sembra essere per le imprese ordinarie

dei consorzi fidi, una realtà tipicamente italiana, che ci mette nelle condizioni di sperare che prima o poi saremo i primi nella logica di una ripresa. Si annoverano inoltre misure urgenti a tutela dell'occupazione:

ai fini della attivazione degli ammortizzatori sociali. Non so quale provvidenza, quale "befana" ci stia dando tutti questi mezzi, però, vero è che questo Governo li ha cercati e trovati. Mai era accaduto che si aprisse la cassa integrazione a tutto Allora ben venga questa azione del Governo e ringraziamo questi uomini che oggi ci stanno dando la gioia di essere all'altezza della situazione. Segue l'attivazione dei fondi per le imprese innovative, per l'intervento nel capitale di rischio e per la capitalizzazione del settore produttivo italiano, che è anemico. Non scordiamoci che rispetto alla Germania, alla Francia ed all'Inghilterra, il bilancio delle nostre aziende per due terzi e è costituito da capitale di terzi e per un terzo soltanto di capitale capitale proprio, quando esiste. Ancora cito l'aiuto al sistema dei trasporti, la disposizione a favore delle piccole e medie imprese, le quote latte. Quanto affetto, signor Ministro, ci lega a voi ed al settentrione ed agli amici delle del settore zootecnico. Sappiamo bene che prestate anche attenzione al settore dell'olio, dei prodotti del Mezzogiorno d'Italia. E apprezziamo l'attenzione che avete riservato alla traslazione del termine dal 31 marzo al 31 dicembre per le agevolazioni previdenziali. È una soluzione che noi ci aspettiamo possa diventare permanente e a regime perché solo così quella solidarietà nazionale, di cui siamo portatori - e ve lo garantisco come uomo che viene da Capo di Leuca - possa germogliare di più anche nei vostri cuori dove sappiamo che già esiste. *(Applausi dal riduzione della spesa pubblica e della pressione fiscale, signori, ho detto all'inizio che non possiamo pretendere di risolvere in queste Aule i problemi che un popolo intero deve e può risolvere come accadde col miracolo italiano. Tutto ciò può accadere soltanto se saremo sempre attenti, unanimemente attenti alla contrazione della spesa pubblica. Per quella via si può sperare in una riduzione della pressione fiscale che sola consente l'elevazione della barca Italia al di sopra di quella che i naviganti chiamano linea di galleggiamento, così da così da metterla nelle condizioni di non essere a livello dell'acqua e di poter navigare per raggiungere porti nuovi e più sicuri. Altri interventi sono per la pianificazione urbanistica: con quanto favore l'Italia guarda a quel provvedimento che il Presidente del Consiglio ha annunciato e che il Governo ha adottato nel cosiddetto piano casa! Questo provvedimento ci libera dai lacci e lacciuoli del nostro apparato pubblico che, pur nella generosità dei lavoratori locali, ha inchiodato il Paese, impedendogli di poter realizzare qualunque iniziativa nel settore della diportistica. E parlo di un settore che per noi che abbiamo le coste che non hanno né la Spagna né la Francia - potrà diventare il settore trainante che solo ci potrà mettere nelle condizioni di produrre beni e servizi laddove esiste la manodopera, sicché la gente possa non emigrare più, da non essere costretti ad erigere monumenti all'emigrante, così come accade o è accaduto in molte parti d'Italia. Allora, signori: fiducia a questo Governo. L'atto di questa sera non è un atto di fede, ma di convinta applicazione delle norme. Guai se non si facesse presto. Facciamo presto, e certamente le istanze e le aspettative che sono anche nei colleghi dell'opposizione, ma che sono in fondo in fondo di tutti gli italiani non saranno disattese.

signori del Governo, onorevoli colleghi, l'attuale scenario economico internazionale sta ponendo nuovi e difficili problemi ai Governi, stretti tra l'esigenza di perseguire una ripresa del ciclo economico, il superamento della crisi finanziaria dei mercati e l'esigenza di mantenere una linea di finanza pubblica rigorosa e lungimirante. In tale contesto, i provvedimenti assunti fino ad ora dal Governo italiano appaiono sicuramente positivi; essi, infatti, sono stati avallati anche dall'Unione europea, la quale ha invece dovuto avviare procedure di infrazione nei confronti di altri Stati membri, che non hanno tenuto in debita considerazione i vincoli comunitari. Di sicuro la crisi internazionale non è ancora cessata, né purtroppo sono certi i tempi di uscita dalla medesima e di ripresa del ciclo produttivo. Permane, quindi, l'esigenza di definire ed attuare ulteriori misure, in favore sia delle imprese che dei lavoratori. Tale esigenza è tanto più profonda in quanto l'attuale crisi non solo è grave, ma è anche lunga, e sono, dunque, messe a dura prova sia la solidità e la vita stessa delle imprese sia la possibilità delle famiglie di riuscire a mantenere un livello di vita accettabile e dignitoso, così come prevede la nostra Carta fondamentale. La fase negativa, peraltro, si innesta in un quadro strutturale che presenta ancora noti problemi, come quello della disuguaglianza tra il Centro Nord ed il Sud del Paese (basti pensare al fatto che, ormai da molti anni, il reddito *pro capite* meridionale non si sposta più da una quota pari al 56 per cento di quello del Centro Nord). L'azione del Governo italiano si sta sviluppando, com'è necessario che sia, lungo diverse direttrici. una ripresa degli investimenti pubblici nelle infrastrutture e nelle grandi opere, in base, in particolare, ai finanziamenti definiti nella seduta del CIPE dello scorso 6 marzo.

all'adozione di una delega per il riordino della disciplina del pubblico impiego, la cui attuazione può determinare il recupero di rilevanti margini di competitività ed un elevamento della qualità dei servizi in favore dei cittadini e delle imprese. infine, un potenziamento degli ammortizzatori sociali, che, come noto facevano parte del collegato alla finanziaria, poi stralciato ed inserito in questo provvedimento, stanti le ragioni di urgenza che giustamente hanno portato a dirottarlo verso questo decreto-legge. questo decreto-legge. A proposito di ammortizzatori sociali, occorre, in primo luogo, sottolineare che la strategia seguita dal Governo è volta a tutelare, al contempo, i lavoratori ed il sistema produttivo, promuovendo, in particolare, il ricorso ad ammortizzatori sociali che non siano automatici e deresponsabilizzanti; la continuità del rapporto di lavoro con le imprese in difficoltà, anche attraverso l'ammissione di proroghe della durata della sospensione, in deroga alla disciplina ordinaria; l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi. in particolare quelle relative all'estensione degli ammortizzatori a categorie di lavoratori fino ad ora sprovviste di tutela, come gli apprendisti e i collaboratori in forma coordinata e continuativa (riguardo a questi ultimi il decreto ha preso in considerazione i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza, i quali sono quelli più assimilabili alla condizione sociale ed economica del lavoratore dipendente); all'introduzione di un indennizzo mensile (fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) per gli esercenti attività commerciali, di età superiore a 62 anni (o a 57 per le donne), in caso di cessazione definitiva dell'attività; alla previsione, in via transitoria, della possibilità di concessione, in favore dei lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'indennità di mobilità, di un trattamento equivalente a quest'ultima. Il decreto n. 185 ha inoltre enunciato in termini generali il principio che ogni trattamento di sostegno al reddito è subordinato - e questo mi sembra un fatto assolutamente nuovo - alla condizione della disponibilità immediata al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. Il combinato disposto dei due provvedimenti costituisce un intervento di grande rilevanza, che consente di attivare risorse pari a 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010 e di sviluppare una politica nel campo degli ammortizzatori sociali improntata sia alla sussidiarietà verticale (tra Stato e Regioni) sia alla sussidiarietà orizzontale (infatti, il decreto n. 185 prevede il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali, in alcuni casi anche subordinando la concessione dei benefici alla condizione di un intervento integrativo da parte degli enti suddetti). Tale linea di intervento è ora sviluppata dal decreto-legge n. 5 in esame, il quale, in materia di ammortizzatori sociali, provvede a semplificare le procedure di concessione del pagamento diretto, da parte dell'INPS, degli interventi di integrazione salariale; a modificare - al fine di adeguarla alle specifiche esigenze dettate da questa crisi - la disciplina per il 2009 della concessione o della proroga di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa ordinaria; a subordinare in via immediata alcune tipologie di indennità di disoccupazione all'intervento integrativo degli enti bilaterali; a raddoppiare, infine, per il 2009, l'importo dell'ammortizzatore sociale per i lavoratori a progetto operanti in regime di monocomittenza.

Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo e sospendo la seduta fino alle ore 19, quando, come preannunciato, avranno inizio le dichiarazioni di voto. *(La seduta, sospesa

Signora Presidente, signori del Governo, il provvedimento in esame e la complessiva vicenda del suo *iter* costituiscono una tappa fondamentale nella definitiva espropriazione del Parlamento e, mi dispiace constatarlo, sanciscono l'assoluta inutilità di questo ramo del Parlamento. In altre parole, si anticipa con i fatti la riforma costituzionale che pone fine al bicameralismo perfetto, trasformando il Senato della Repubblica in un organo dal carattere meramente consultivo. Questa affermazione poggia su dati di fatto inoppugnabili. In primo luogo, il decreto-legge giace da quasi due mesi alla Camera, dove è stato approvato con l'apposizione della fiducia, e il Senato è costretto, sempre con la fiducia, ad approvarlo in due giorni, pena la decadenza del decreto-legge stesso. Ciò si traduce non solo nell'impossibilità di garantire il dettato costituzionale, ma anche nel disattendere l'attuale Regolamento del Senato che prescrive per l'approvazione dei provvedimenti un attento esame e un'ampia discussione, sia in Commissione sia in Aula.

Sembra quasi di assistere al gioco delle tre carte, il gioco che serve ad ingannare i gonzi, senza considerare la più seria obiezione della mancanza di copertura del provvedimento sulle quote latte che ne mette in pericolo la promulgazione. Ricordiamo, inoltre, che con quel decreto-legge gli allevatori del Mezzogiorno, che si sono comportati virtuosamente e nel rispetto dei vincoli, sono costretti a subire i comportamenti scorretti di taluni allevatori del Nord, cosa di cui il Governo mena gran vanto. Faccio poi riferimento, nel merito del provvedimento, ad un punto per noi essenziale relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. Già con il maxiemendamento oggetto della fiducia, in cui si inseriscono le norme relative all'assegnazione delle quote latte

Ma la perla di questo decreto-legge è lo sconsiderato saccheggio della quota dei fondi previsti vincolati al sostegno e al rilancio delle aree meridionali. Si tratta di un vero e proprio "riciclaggio di risorse" al quale si procede attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge anticrisi dello scorso anno che interveniva sul criterio di ripartizione territoriale delle risorse, richiamando esplicitamente il vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del 15 per cento Si introduce sostanzialmente un meccanismo che consente la "pulizia" di risorse che possiedono un obbligo di impegno e di distribuzione territoriale, sancito dalla legge istitutiva del FAS che, una volta stanziate e non ancora impegnate dalle Regioni o dallo Stato,

stabiliti dall'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza alcun vincolo territoriale,

A questo punto una domanda sorge spontanea. A chi andranno queste risorse? Quale sarà la loro destinazione? Verrà avvantaggiata ancora una parte del Paese e sarà ancora il Sud Quel Sud, ricordiamolo, sottosviluppato che, oltre ad essere stato sempre penalizzato e non sufficientemente sostenuto in passato, deve ora affrontare una gravissima crisi economica, che è crisi anche per noi, con un sistema produttivo, infrastrutturale e sociale debolissimo, senza adeguata attenzione da parte del Governo che continua a non offrire risposte soddisfacenti alle richieste di quest'area del Paese alla quale, sin dall'inizio della legislatura, ha deliberatamente sottratto e tagliato cospicue risorse economiche.

Per non parlare delle risorse del FAS, quota regionale, ancora formalmente attribuite alle Regioni del Sud, ma alle stesse, nella sostanza, non destinate dal CIPE, malgrado l'istruttoria completata positivamente dal Ministero dello sviluppo economico, competente per materia. Parliamo, per esempio, delle risorse del POR Sicilia, deliberate dal CIPE il 6 marzo, che ancora sono ferme e non vengono destinate. Ma il saccheggio delle risorse destinate prioritariamente al Mezzogiorno non finisce qui. Nel decreto-legge che stiamo per votare sono ancora ingenti le risorse stornate: 400 milioni di euro per il 2009, da utilizzare

ma è divertente pensare che perfino l'ulteriore finanziamento dell'operazione Alitalia viene pagata con fondi del FAS. Si istituisce, inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, un nuovo fondo, denominato "Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale" che diventa destinatario delle risorse FAS, che ammontano a circa 9 miliardi di euro (delibera CIPE del 6 marzo). Cosa nasconde l'istituzione di questo nuovo Fondo, che sembrerebbe una operazione di semplice *maquillage*, mentre in realtà il provvedimento non prevede nulla riguardo alla destinazione, all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse il cui utilizzo, mi dicono, è svincolato da qualsiasi programmazione, ma funziona discrezionalmente, a domanda, come uno sportello bancario privato? In questa prima fase di legislatura, il Movimento per l'Autonomia si è impegnato in un'azione parlamentare molto forte con la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al fine di difendere il criterio di ripartizione Nord-Sud previsto dalla legge, avendo colto nell'azione del Governo una costante attitudine a utilizzare le risorse destinate al Mezzogiorno per fini, magari, di sostegno reale dell'economia nazionale nel suo complesso, in questa fase di crisi economica generale. In sintesi, come nel 1860 l'Unità nazionale si finanziò con i soldi depredati al Sud e nel dopoguerra il processo di industrializzazione del Paese fu realizzato attraverso la migrazione forzata della forza-lavoro del Mezzogiorno, oggi si fronteggia la crisi economica di quel sistema finanziario, tutto allocato al Centro-Nord, con le risorse che erano destinate, sulla carta, a promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali. Il Governo più volte si è impegnato a recepire le sollecitazioni e le proposte che provenivano dal nostro Movimento, accogliendo ordini del giorno o introducendo esplicitamente nelle norme di legge il criterio di ripartizione che, a nostro avviso, sarebbe risultato ultroneo, stante il vincolo preciso insito nell'istituzione dei Fondi Il principio generale della legislazione, però, per cui una legge successiva modifica quella precedente, vanifica di fatto questo criterio di ripartizione; attribuendo al Governo, che per legge preleva le risorse - e lo può fare, ovviamente un potere assoluto e discrezionale nell'utilizzo di queste stesse risorse, anche perché dobbiamo prendere atto dell'impotenza assoluta del Parlamento ad incidere sugli atti predisposti dal Governo. Di fronte a tutto questo il comportamento naturale sarebbe quello di far prevalere la passione di parte e la voglia di affermare con forza le ragioni del nostro radicamento territoriale negando la fiducia al Governo su questo provvedimento, della ineluttabilità di questo Esecutivo, al quale il Paese, e il Mezzogiorno in particolare, ha affidato la propria aspettativa di benessere e di serena convivenza civile, che in questa fase così drammatica assume un valore quasi ultimativo, ci inducono a sperare in un ravvedimento profondo nell'azione di governo che sappia finalmente rispondere, con equità, agli interessi di tutta la comunità nazionale superando questa politica strabica. Per questa speranza, oltre che per la coerenza sempre confermata al patto elettorale e politico sancito con gli elettori, confermo ancora una volta, con fatica, la fiducia al Governo della Repubblica.

provvedimento che, fino a poco tempo fa, recava solo misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e che oggi viene integrato con il nuovo tema, assai controverso, delle quote latte. Il Governo ci stupisce ogni giorno di più, riesce sempre a trovare una nuova forzatura, un modo diverso per eludere il Parlamento, per infilare qua e là provvedimenti che nulla hanno a che vedere con la materia in esame. La capriola legislativa questa volta ha dell'incredibile: si è inserito parte di un decreto-legge non convertito in un altro decreto‑legge, e lo si è fatto in sede di conversione, oltretutto ricorrendo al voto di fiducia. Assistiamo ormai, cari colleghi, ad un balletto di norme degno del migliore Bolshoi, a cui il Parlamento, sordo e grigio, è tenuto a fare da pallido spettatore.

ciò che è avvenuto alla Camera, ossia l'aver trasposto in un altro provvedimento le norme che riguardano le cosiddette quote latte e che disciplinano l'assegnazione del quantitativo nazionale garantito di latte, nonché la rateizzazione dei debiti contratti dagli allevatori relativamente alle cosiddette quote latte. Si sono inserite tali disposizioni del tutto estranee rispetto alla materia disciplinata dal decreto-legge oggetto di conversione, che incidono in ambiti materiali diversi e per cui non sussistono adeguate ragioni di necessità ed urgenza. In altri termini, appare evidente che eventuali ragioni di urgenza riferite alla crisi di alcuni settori industriali non possono giustificare interventi a sostegno degli allevatori. Su questo punto, cari colleghi, la sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 2007 è estremamente chiara. La Corte ha sottolineato che «la legge di conversione di un decreto‑legge è caratterizzata nel suo percorso parlamentare da una situazione tutta particolare, al punto che la presentazione del decreto-legge per la conversione comporta che le Camere vengano convocate ancorché sciolte (...), e il suo percorso di formazione ha una disciplina diversa da quella che regola l'*iter* dei disegni di legge proposti dal Governo». Quindi, non solo ci troviamo nel caso della carenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, con riferimento agli articoli 8-*bis* e seguenti inseriti surrettiziamente nel disegno di legge di conversione del decreto‑legge, ma ci troviamo di fronte all'ipotesi ancora più grave di surrettizia violazione del divieto di reitera dei decreti-legge, tenuto conto del fatto che il testo del decreto-legge non convertito risulta trasposto nel disegno di legge di conversione di altro decreto-legge.

È una vera e propria vergogna ed è una vergogna istituzionale. Tralascio i profili evidenti di violazione dell'articolo 3 della Costituzione e la circostanza che state mortificando gli allevatori perbene. Proprio per questa ragione, vorrei farvi presente che, al di là del metodo eccessivamente creativo che avete seguito, è soprattutto il merito che ci preoccupa, perché il fulcro di questo provvedimento è finito per diventare proprio il decreto-legge sulle quote latte, che era stato ragionevolmente accantonato, viste anche le proteste degli allevatori in piazza. Ora questo testo ha solo un significato politico: dare un po' di ristoro ai colleghi della Lega Nord, che peraltro oggi alla Camera sono usciti sconfitti politicamente su altri temi. In realtà, coloro che in questi anni hanno violato sistematicamente le norme nazionali e comunitarie, splafonando e rifiutandosi di pagare, vengono premiati con una sanatoria, mentre la stragrande maggioranza degli allevatori onesti con sacrifici ha sempre pagato tutto, scegliendo di operare nel pieno rispetto delle regole: una disparità di trattamento rispetto a chi ha limitato i propri investimenti, ha tirato la cinghia in un periodo di crisi economica, pur di adeguarsi alle norme comunitarie. decreto-legge in discussione suona come uno sberleffo, come un'istigazione a far parte anche loro della casta cosiddetta dei "furbetti del latticino". Altro che libera concorrenza, altro che libero mercato e sussidi all'industria dell'auto! Siamo ai sussidi di illegalità, altra categoria mirabilmente inventata da questo Governo. All'interno di questo provvedimento ci sono una serie di iniziative anticrisi che noi abbiamo valutato senza pregiudizi e con attenzione, vista la gravità della situazione economica del nostro Paese. Mi riferisco agli ecoincentivi, agli incentivi per la rottamazione delle vecchie vetture e degli elettrodomestici. Ci troviamo, però, sempre di fronte a toppe, a piccoli interventi, che non riescono tutti insieme a rispondere alla crisi e che forse potrebbero anche rivelarsi negativi nel medio e nel lungo periodo, se si pensa che i provvedimenti che riguardano il settore dell'auto si inquadrano in una logica protezionistica europea che non fa bene al mercato e che sottrae risorse a sostegno di settori in cui il mercato non è saturo.

D'ALIA). Valutiamo positivamente il principio in forza del quale i Comuni virtuosi possono aumentare le spese per la sicurezza e gli interventi sociali, anche se il limite di 150 milioni di euro ci appare troppo stringente.

e quindi fa un'attività d'impresa, e chi delocalizza con il solo obiettivo di speculare sul costo del lavoro. Non crediamo poi, signor Presidente, che il sostegno alle fasce deboli possa concretizzarsi - con tutto il rispetto - con un *decoder* digitale in più o in meno. Sarebbe stato meglio forse garantire sostegni al reddito e assicurare maggiori servizi, compresa una politica sui prezzi che passi dall'abbattimento di quelle rendite che sono oggi i servizi pubblici locali, gestiti in situazione di monopolio, che determinano

utilizzati sempre più per coprire interventi che con lo sviluppo delle aree depresse non hanno alcun legame. Sarebbe stato più onesto, visto che parliamo di sostegno al settore dell'auto,

umiliazione della sottrazione di fondi rispetto alle loro finalità di istituto. Poi ci siamo inventati la copertura da "furbetti del quartierino" con l'impiego

poiché ha mostrato preoccupazione, anche se non ha azzardato soluzioni adeguate e credibili, anzi, prima ha annunciato di essere pronto a sforare ulteriormente il rapporto deficit/PIL... finanziando in deficit le politiche anticrisi, poi ha smentito lasciando tutti perplessi. Siamo alle solite: si alza il tono di voce, ma non si alza il livello degli interventi contro la crisi. Siamo convinti che da questa spirale negativa si possa uscire, ma solo con un insieme di riforme organiche, poche, coraggiose, forse anche un po' impopolari, che abbassino magari le percentuali di qualche sondaggio, ma che possano davvero provocare un'inversione di tendenza, a partire dalla riforma delle pensioni, il sostegno al reddito delle famiglie e delle piccole e medie imprese, con una legislazione bancaria più trasparente nell'erogazione del credito e nel rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese e con una riforma contro gli sprechi e le inefficienze della pubblica amministrazione. Fino ad oggi, signor Presidente, abbiamo visto solo promesse, affrettate smentite e interventi parziali, dislocati in tanti diversi calderoni di norme, senza mai una visione d'insieme. In altre parole, ci troviamo di fronte ad una terapia medica che somministra l'aspirina per curare la polmonite. In questo decreto-legge, in particolare, i già pochi e deboli provvedimenti contro la crisi vengono oscurati dall'arroganza delle quote latte, rendendo questo testo invotabile e indigeribile, come il latte che il Governo ha mandato di traverso agli allevatori perbene. Votiamo no alla fiducia e a questo provvedimento poco serio e inutile. Quando ci porterete provvedimenti buoni, ve li voteremo. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anzitutto mi sia consentito di esprimere il cordoglio più sincero per le vittime del terremoto che ha devastato L'Aquila e e altri paesi del vicino Abruzzo. Una tragedia che ha colpito la nostra terra. Assieme al senatore Mascitelli siamo stati in queste ore ad Onna, un paese distrutto, letteralmente raso al suolo dal sisma che ha seppellito sotto le macerie molti bambini. Anche noi associamo la nostra gratitudine alla macchina della Protezione civile, ai carabinieri, ai poliziotti, ai soldati, vigili del fuoco, alla Guardia di finanza, ai militari, al Corpo degli alpini, al mondo del volontariato e a tutti coloro che si sono prodigati, fin dal primo momento, per portare sollievo alla popolazione duramente colpita da una immane tragedia. Ma dopo aver visitato l'ospedale da campo, allestito accanto all'ospedale costruito soltanto pochi anni fa, probabilmente al di fuori delle normative antisismiche, mi preme portare alla sua attenzione, signor Presidente del Senato, mi preme portare alla sua attenzione, signor Presidente del Senato, affinché lei possa esprimerle al Governo, le richieste dei medici e degli infermieri che si stanno prodigando notte e giorno per assistere gli ammalati ed i feriti. Mancano i *container* ed i camper per i medici, per dare loro la possibilità di cambiarsi, lavarsi e riposarsi. Formuliamo queste richieste, signor Presidente, senza alcuno spirito polemico, augurandoci che possano essere accolte. È difficile, dopo aver visto con i nostri occhi il dolore composto di tanti conterranei che hanno perso i loro cari,

recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, inizialmente finalizzato a fronteggiare la crisi internazionale del settore industriale, con particolare riferimento al comparto automobilistico, anche in relazione alle implicazioni sul sistema produttivo nazionale e ai riflessi di carattere occupazionale

antiparlamentare del Governo; inoltre, a seguito della presentazione del maxiemendamento, risulta oggi ulteriormente integrato con le norme contenute nel decreto-legge sulle inevitabilmente, che il provvedimento reca un contenuto alquanto disomogeneo, che spazia dalla rottamazione di auto e moto al finanziamento del fondo di garanzia per le imprese, passando per i microrimborsi per i risparmiatori Alitalia. Non diciamo che è tutto da buttare. Ci sono luci ed ombre, ma ci sono più ombre che luci in questo provvedimento, mi riferisco soprattutto ad alcuni articoli. Il Gruppo dell'Italia dei Valori, già in sede di discussione alla Camera dei deputati, aveva espresso la sua netta contrarietà alla richiesta del voto fiducia su questo provvedimento, motivando ragioni di merito e metodo che non voglio replicare. Pertanto, non potremo esprimere un voto favorevole per alcuni ragioni che passo ad elencare: anzitutto l'articolo 5-*bis*, probabilmente incostituzionale, con il quale si riducono i vincoli per la conversione di vecchie centrali elettriche inquinanti inquinanti in nuove strutture a carbone, come ad esempio la centrale di Porto Tolle. In particolare, la norma in questione prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge

Nord. Ci apprestiamo ad approvare il federalismo fiscale, eppure alcuni provvedimenti vanno contro l'autonomia delle Regioni. Mi riferisco alla legge regionale n. 1997, istitutiva del Parco regionale del Delta del Po, che vieta l'insediamento di centrali a combustibili più inquinanti del gas metano.

Oltre a ciò, vorrei ricordare anche le ragioni che inducono l'Italia dei valori a votare Un'altra ragione l'ha ricordata anche il presidente D'Alia: mi riferisco al pozzo di San Patrizio dei fondi dormienti delle banche che dovrebbe finanziare gli obbligazionisti e i risparmiatori che sono stati truffati dai *bond* argentini, ma soprattutto quelli di Alitalia. Il Governo ha affermato che l'offerta presentata da CAI-Compagnia aerea italiana S.p.A, in data 31 ottobre, per l'acquisto di complessi di beni e contratti del gruppo Alitalia, non prevede l'emissione, da parte di CAI, di *warrant* da scambiare con azioni o obbligazioni Alitalia. Tra l'altro,

cento 2002-2010 convertibile», emesso da Alitalia linee aree italiane, ora in amministrazione straordinaria, il diritto di cedere tale obbligazione al Ministero dell'economia e delle finanze in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012. Agli oneri derivanti da questa disposizione, nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse provenienti da questo pozzo di San Patrizio dei conti dormienti. Già mi sono soffermato su questo, come sui "Mengozzi *bond*" e quindi sulla difficoltà di rimborsare gli obbligazionisti. Il Governo, in risposta ad un'interrogazione presentata presso la 6a Commissione permanente della Camera dei deputati, il 22 gennaio ha dichiarato in che modo intende rispettare l'impegno di tutelare gli oltre 40.000 sottoscrittori del prestito obbligazionario, ossia i "Mengozzi *bond*"*.* Nel decreto ci sono anche misure condivisibili, come quelle previste dall'articolo 7-*ter* a tutela dell'occupazione, il pagamento diretto ai lavoratori contestualmente all'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fatta salva la revoca in caso di assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa, il raddoppio dell'indennità di disoccupazione dal 10 al 20 per cento per i co.co. pro., che restano senza lavoro, e la possibilità per chi beneficia di una forma di ammortizzatore sociale di svolgere anche piccoli lavori a pagamento senza perdere l'assegno. essendovi più ombre che luci in questo provvedimento (che se non fosse stata posta la fiducia l'opposizione avrebbe potuto contribuire a migliorare) essendo stata posta l'ennesima fiducia, l'Italia dei Valori non potrà che votare contro un decreto tardivo, che poteva essere migliorato dal contributo responsabile dell'opposizione. Per queste ragioni, ripeto, non possiamo votare la fiducia al Governo. *(Applausi dal

Ci troviamo oggi a votare in fretta due decreti-legge e li voteremo insieme perché gli stessi, se fossero decaduti, avrebbero procurato a questo Paese effetti disastrosi. Di questo siamo convinti. Le misure adottate dal Governo per affrontare la crisi economica rientrano in un quadro più generale di interventi che da tempo sono stati messi in campo attraverso l'adozione di diversi decreti tra di loro strettamente collegati. Si tratta, in realtà, di misure che hanno origine a partire dalla anticipazione della manovra finanziaria dell'estate scorsa e che proseguiranno, al di là dell'approvazione del presente decreto, avendo come fine ultimo di sostenere le imprese e le famiglie in questo momento difficile e restituire a questo Paese nuove prospettive di crescita. La crisi economica in atto nel Paese sta letteralmente paralizzando il sistema produttivo, impedendo alle piccole e medie imprese di crescere ed essere maggiormente competitive sul mercato. La strada intrapresa ha quindi portato all'adozione di un pacchetto di aiuti che, inizialmente rivolti a sostegno di settori mirati, primo tra tutti quello automobilistico, sono stati poi estesi ad altri settori comunque colpiti dalla crisi economica. Il testo in esame conferma quindi gli incentivi varati d'urgenza dal Governo per l'acquisto di veicoli, mobili ed elettrodomestici, lasciando poi però spazio ad altre importanti misure a tutela delle imprese nazionali. Anche il settore tessile, come peraltro da noi della Lega Nord fortemente auspicato, ha trovato spazio all'interno del provvedimento, attraverso l'assegnazione diretta di risorse che interesseranno anche i settori della concia e calzaturiero, risorse assegnate solo a quelle aziende che hanno trovato soluzione per gli scarichi industriali e che saranno effettive solo dopo l'emanazione di specifici decreti attuativi. attuativi. Siamo convinti che le misure del presente decreto siano necessarie ed importanti per affrontare la crisi. Tuttavia, non possiamo permetterci ritardi nella realizzazione degli interventi prospettati, soprattutto a tutela delle imprese nazionali. Vorrei ricordare, infatti, che accanto ai grandi colossi industriali esiste una realtà fatta di tante piccole e medie imprese che non possono essere dimenticate, dal momento che rappresentano il punto di forza di tutto il sistema produttivo nazionale. Questa è una realtà per anni ignorata, ora scoperta e rivalutata dalla stessa Comunità europea, che nello *Small Business Act* non solo ne riconosce l'indispensabilità, ma detta un decalogo per incentivarne la nascita e lo sviluppo.

solo attraverso le piccole e medie imprese e le piccole banche territoriali. Noi l'avevamo sempre detto e sostenuto: la Lega Nord ha sempre professato questo tipo di posizione in favore delle piccole e medie imprese e delle banche territoriali. Purtroppo, però, queste imprese stanno attraversando una fase assolutamente critica, che ha pesanti ripercussioni in termini occupazionali. È pertanto fondamentale salvaguardare tali realtà produttive, che rappresentano un grande bacino di ricchezza per il Paese, le cui potenzialità tuttavia devono essere sfruttate al meglio per garantire il costante e duraturo sviluppo economico dei nostri territori. Come ha sempre sostenuto la Lega Nord, solo una maggiore attenzione al territorio e alle sue risorse umane e produttive può risolvere la crisi. In questo contesto, riteniamo fondamentale che il Governo, accogliendo un'istanza del nostro Gruppo, sia riuscito a imporre il divieto per le aziende di delocalizzare le attività produttive al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo,

che lo Stato riconosca aiuti a quelle aziende che magari, una volta ottenuti i vantaggi per loro, portano la produzione all'estero, creando disoccupazione nel nostro territorio. Avremmo preferito approfondire, durante l'esame in Aula, le problematiche prima richiamate, al fine di dare maggiore correttezza alle misure adottate per tutelare le imprese e l'occupazione, ma ciò non è stato possibile, per i tempi ristretti che abbiamo a disposizione. Ci auguriamo pertanto che nei successivi provvedimenti il Governo voglia dedicare maggiore attenzione alle proposte che vanno nella direzione indicata dalla Lega Nord. Siamo convinti che si stia facendo il possibile, anche alla luce delle poche risorse disponibili, per uscire dalla crisi e riportare il Paese su più alti livelli competitivi. Le basi esistono, sono concrete. Aspettiamo soltanto di poter raccogliere nel più breve tempo possibile i frutti delle misure fino ad oggi messe in campo per sostenere la ripresa economica del Paese.

Ma, come ha ben esplicitato il collega Vallardi nel suo intervento, ciò che è importante è la serenità delle famiglie dei lavoratori e produttori del mondo agricolo, che hanno bisogno più che mai di essere tutelate, difese, per continuare a produrre quei prodotti di qualità e di eccellenza di cui tanto andiamo fieri. gente che svolge una professione dura, fatta di sacrifici, poche soddisfazioni e che grazie a questo Governo e al nostro ministro Zaia, che ringraziamo, inizia ad intravedere la via del rilancio e di una nuova considerazione.

Signor Presidente, trovo che sia particolarmente difficile per ciascuno di noi superare il senso di pochezza di queste discussioni, a fronte della tragedia che numerosi cittadini italiani stanno vivendo a L'Aquila e nei territori così gravemente colpiti dal terremoto. Chi non è interessato all'intervento del senatore Bubbico è pregato di lasciare l'Aula, dopo un minuto si tornasse allo *status quo ante*.

che mettono a nudo la fragilità della nostra ostentata sicurezza, alimentata spesso da pensieri brevi e sbrigativi. Conosciamo, come popolo italiano, io credo, i nostri vizi, ma abbiamo a disposizione anche i buoni esempi, rappresentati dai risultati conseguiti, quando decidiamo di mettere in campo le nostre migliori virtù. E l'Italia, nel corso degli anni, ha saputo superare momenti difficili; ha saputo raggiungere traguardi importanti quando non si è cullata nella convinzione che poi tutto si aggiusta o che altri possano pensare per noi. In questo disegno di legge, signor Presidente, quello che ci appare più rilevante è proprio la carenza di un'idea, di un progetto, di una tensione rispetto alle sfide importanti. Eppure siamo al sesto intervento contro la crisi. E sembra quasi che ogni volta si sbaglino i tempi e i modi. Si vanificano le procedure già avviate, già mature per promuovere attività e cantieri nell'intento di concentrare le risorse su pochi grandi obiettivi strategici, la cui cantierabilità viene rinviata nel tempo per poi ritornare sui propri passi e accorgersi che invece è necessario mettere in campo l'operatività del nostro Paese, in grado di promuovere tutte le opportunità derivanti dalla capacità di fare sistema. Si interviene deprimendo la domanda pubblica e privata, quando invece sarebbe necessario sostenerla e si presume di aiutare le imprese a produrre di più quando si consuma di meno. Queste sono contraddizioni evidenti nei ragionamenti che non abbiamo potuto sviluppare nei tempi giusti in questa circostanza. Si rinuncia, quindi, a pronunciare e a sostenere investimenti strategici sulla ricerca e sullo sviluppo per attrezzarsi ad affrontare le nuove sfide competitive, quelle che risulteranno ben più complesse quando il ciclo cambierà. è una qualche relazione tra quanto si sta facendo nel nostro Paese e quanto si sta facendo nel resto del mondo? Io credo che non ci sia nessuna relazione. Si pensa di affidare l'efficacia delle misure alla *moral suasion*; si pensa di premiare le aziende che non delocalizzano, quando invece siamo di fronte ad una profonda crisi di domanda, quando siamo di fronte ad una crisi di fiducia da parte dei cittadini. Voglio aggiungere, signor Presidente, che in una situazione di difficoltà è semplice eccepire che quanto viene proposto o quanto viene fatto è insufficiente o inutile o addirittura sbagliato. Ma non è questo lo spirito con il quale abbiamo lavorato in queste poche ore di confronto che ci sono state concesse dalla decisione del Governo di chiedere il voto di fiducia. Non è questo il senso dei numerosi e qualificati interventi pronunciati in quest'Aula dai tanti senatori del Partito Democratico, interventi carichi di proposte, di sensatezza, di azioni definite perché si possa superare la crisi. crisi che temiamo sarà più lunga di quanto si pensi e le misure varate con questo provvedimento non saranno sufficienti - ne siamo certi - a farvi fronte. quindi a discutere di crisi e di misure a sostegno dei cittadini e delle imprese e vorremmo annunciare sin d'ora il nostro auspicio...

quel senso dell'interesse generale e quella mobilitazione in grado di chiamare tutti ad esercitare la propria responsabilità e ad offrire il proprio contributo. Esattamente come hanno fatto le Regioni, quelle meridionali in modo particolare, quando hanno messo a disposizione le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, rinunciando anche al riparto dell'85 per per dotare il Fondo per gli ammortizzatori sociali, che risultava privo di risorse finanziarie. Ma quella abnegazione, quell'attenzione, quella cura dell'interesse generale ci sembra non venga sufficientemente colta da parte del Governo perché si pensa che il dialogo, il confronto, la condivisione non servano. Questo è sicuramente il più grave dei difetti insiti in tale provvedimento, come in tutta la condotta del Governo. Abbiamo l'impressione che si agisca alla ricerca di nuovi strumenti da comunicare e da far vivere giusto fino all'annuncio di strumenti successivi, com'è accaduto con i provvedimenti varati quando, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, furono costituite ed assegnate le risorse relative a progetti non ancora cantierizzati

è poi proceduto a modificare quella decisione; con questo provvedimento si prelevano infatti le risorse già assegnate al Fondo per la competitività e lo sviluppo e le si mettono a disposizione del Fondo strategico per il Paese, a sostegno dell'economia reale, quasi che la competizione, lo sviluppo, la ricerca e l'innovazione non fossero economia reale. Nel frattempo, lo spostamento di risorse dal Fondo per la competitività al Fondo strategico per il Paese si perdono per strada 600-700 milioni di euro, 400 dei quali vengono messi a disposizione di interventi connessi ad eventi celebrativi, di cui c'è pure necessità e bisogno ma che non ci sembra meritino la mobilitazione di risorse destinate invece a promuovere quella spinta in avanti di cui il Paese ha tanto bisogno. Ci sono poi le questioni relative alle scelte compiute in questa circostanza ponendo la fiducia su un provvedimento le cui criticità sono state segnalate dalle organizzazioni agricole e poi riprese in quest'Aula. ne sono di questioni sulle quali riflettere, signor Presidente. Ci sarebbe e c'è tanto da fare e il Partito Democratico è pronto a dare il proprio contributo per il Paese e per i nostri cittadini in difficoltà,

ma vorremmo tanto poter votare a favore di un provvedimento a sostegno delle azioni necessarie per rilanciare il nostro Paese. Grazie, Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge all'esame del Senato costituisce uno dei principali provvedimenti

scusi, senatrice Vicari. Colleghi, siamo alla fine di questa seduta, ma non intendo proseguire i lavori con questo brusìo. Scusate, ma sarò costretto tra poco ad interrompere i lavori, così ritarderete tutti di un'ora l'arrivo a casa. Ho 30 richieste di voto anticipato sulla fiducia: c'è tanta fretta di concludere questi lavori, ma non c'è la volontà di farlo con compostezza.

Il provvedimento d'urgenza, infatti, costituisce l'ultima delle misure varate dall'Esecutivo che, fin dall'inizio della crisi, è intervenuto con vigore per tutelare prima di tutto i risparmiatori; per evitare strette creditizie alle imprese e alle famiglie; per rilanciare i consumi; e, soprattutto, per dare nuova fiducia agli italiani. L'esame del provvedimento da parte del Senato avviene purtroppo in un momento particolarmente drammatico per la storia del nostro Paese, a seguito del terremoto che ha colpito in maniera così violenta la Regione Abruzzo. A questo proposito, consentitemi una doverosa digressione, che però rafforza il peso di quanto questo provvedimento contiene, perché alle popolazioni delle zone colpite dal sisma deve andare sì in questo momento la nostra solidarietà, ma, soprattutto, un messaggio di fiducia e di speranza. Tale fiducia dovrà essere alimentata dalla certezza di una ricostruzione nei tempi più rapidi possibili. Il Governo infatti, dopo aver immediatamente seguito le operazioni di soccorso, fin dalle prime ore, sta ora lavorando ad un pacchetto di aiuti economici immediati, il cui obiettivo sarà di dare, appunto, nuova speranza alle popolazioni colpite dal Per affrontare la crisi economica, invece, altrettanta fiducia deve essere trasmessa alle famiglie italiane. Il decreto-legge anticrisi si muove in questa direzione, attraverso un rilancio prima di tutto dei consumi: ecco il perché, ad esempio, dell'introduzione di appositi incentivi per il settore dell'auto, che da sempre costituisce un comparto fondamentale dell'economia nazionale. Gli incentivi varati dal nostro Governo non costituiscono un aiuto pubblico alle imprese, come avvenuto invece in Francia, dove consistenti risorse sono state dirottate a favore dei grandi colossi dell'auto. Noi, nell'ottica di mettere al primo posto le famiglie, abbiamo previsto degli incentivi per promuovere il consumo diretto di beni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. I *bonus* per la rottamazione auto hanno consentito, nel mese di marzo, di raddoppiare le immatricolazioni e di far ripartire questo settore. Le misure varate stanno consentendo di rinnovare il parco auto italiano, particolarmente vecchio e quindi inquinante, e di garantire al Paese il pieno rispetto degli impegni assunti nelle sedi internazionali, a partire proprio dal pacchetto clima-energia, approvato nel dicembre scorso. Gli incentivi statali cumulabili con le misure che alcune Regioni italiane hanno adottato, consentono ora ad una famiglia media di acquistare un'auto ecologica a metà del prezzo che avrebbe pagato solamente due mesi fa. Agli incentivi per il settore dell'auto si aggiungono poi i*bonus* per gli acquisti di elettrodomestici. Anche in questo caso il Governo ha ritenuto di promuovere i consumi delle famiglie italiane verso l'acquisto di prodotti che garantiscono un maggior risparmio energetico. La vendita di questi prodotti sta già assicurando, ad un settore in crisi come quello del bianco, nuove possibilità per un rilancio complessivo. Gli incentivi legati alla ristrutturazione degli immobili si intersecano con la prossima approvazione del piano casa, che consentirà di rimettere in moto anche il comparto dell'edilizia. I dati ci dicono che, se soltanto il 10 per cento delle famiglie italiane decidesse di procedere a ristrutturazioni ed ampliamenti della propria abitazione, verrebbero subito messi in circolazione circa 60 miliardi di euro. Si è poi prestata particolare attenzione al mondo delle imprese che, insieme alle famiglie italiane, consentiranno all'Italia di superare in tempi brevi la crisi economica. Ci tengo a ricordare la disponibilità del Governo e del presidente del Consiglio Berlusconi in particolare a comprendere subito le istanze provenienti dal mondo imprenditoriale, attraverso un confronto proficuo con la presidente di Confindustria Marcegaglia. Il provvedimento al nostro esame ha recepito le richieste pervenute dal mondo imprenditoriale e gli accordi raggiunti con le diverse categorie nei tavoli tecnici presso il Ministero dello sviluppo economico. Pertanto, colleghi, sono prive di fondamento le considerazioni di coloro che nella giornata di oggi hanno dichiarato che le istanze del mondo imprenditoriale non sono state attentamente valutate dal Governo e che i problemi delle associazioni audite dalle Commissioni parlamentari non hanno trovato alcuna risposta. Tutto il contrario, colleghi. Il decreto, invece, ha previsto una serie di importanti agevolazioni fiscali volte a favorire le aggregazioni di imprese e la ristrutturazione delle stesse, le reti di imprese e i distretti industriali. Gli imprenditori italiani potranno contare, inoltre, su un Fondo di garanzia particolarmente cospicuo. Il decreto, infatti, mette a disposizione più di un miliardo di euro per l'accesso al credito delle imprese. Come è stato autorevolmente detto, il mondo bancario non potrà ora più negare alle imprese sane il credito di cui hanno bisogno per programmare i propri investimenti.

Grazie, signor Presidente. Abbiamo inoltre prestato attenzione ad alcuni specifici settori, come quello tessile e calzaturiero, prevedendo, anche in questo caso, un Fondo di garanzia specifico. Particolare sensibilità è stata dimostrata nei confronti del mondo del lavoro e dei lavoratori precari. La semplificazione delle procedure per l'ottenimento della cassa integrazione consentirà una sensibile riduzione dei giorni necessari all'erogazione degli ammortizzatori sociali. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge sul quale il Senato si appresta oggi a dare la propria fiducia costituisce una tessera fondamentale del mosaico dell'intera azione che l'Esecutivo ha messo in atto per affrontare la crisi economica. Nessuno nega che la crisi esista in Italia come negli altri Paesi dell'Unione europea e non solo e nessuno vuole negare le ripercussioni che questa crisi sta avendo sulla società. Il Governo sta affrontando seriamente ed in maniera determinata una crisi planetaria che somma come suo effetto vecchie e nuove povertà. La risposta a questa crisi deve essere globale e infatti noi stiamo proponendo soluzioni che puntano a sostenere il più possibile il mercato interno e che sono già state condivise a livello comunitario nonché dagli altri Paesi del G8. Le misure previste fino ad ora sono volte a: sostenere i redditi; tenere alta la domanda interna per non far flettere la produzione; ammodernare le strutture dello Stato. In quest'ottica noi puntiamo: alla produzione di ricchezza e di lavoro; a sostenere le piccole e medie imprese; a una pubblica amministrazione efficiente e capace di rispondere in tempo reale alle esigenze di sviluppo della nostra società. Per questo il PdL darà con convinzione il voto di fiducia al Governo, per sostenerlo nella sua azione complessiva contro la crisi e la recessione, rispettando il mandato ricevuto da milioni di italiani che, con il voto a Silvio Berlusconi ed al Popolo della Libertà, hanno dato fiducia a questa politica e a queste scelte per un futuro di ripresa e di crescita nell'interesse del popolo italiano. orgogliosi di avere assicurato, con importanti incentivi, la ripresa dei consumi; noi siamo orgogliosi di aver favorito le aggregazioni d'impresa; noi siamo orgogliosi di avere puntato sui distretti industriali e sulle reti di imprese e di aver premiato, con riguardo al Patto di stabilità, le amministrazioni locali virtuose; noi siamo orgogliosi di aver assicurato ai lavoratori precari un robusto sistema di ammortizzatori sociali; ma, soprattutto, siamo orgogliosi di avere dato, con i provvedimenti finora varati, un'iniezione di fiducia a tutti gli italiani. Quella fiducia e quella speranza che si sta diffondendo nel Paese e che consentirà ancora una volta di superare tutte le difficoltà.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

i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Poiché 29 senatori hanno chiesto di anticipare il voto rispetto all'ordine della chiama, la Presidenza ritiene opportuno, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori,

Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora,

non l'hanno firmata in questo momento) di verificare con il Governo le modalità per utilizzare il montepremi del Superenalotto a favore dei terremotati.

che può dare il senso di quella solidarietà nazionale che stiamo cercando tutti di costruire intorno a tale evento e che magari anche le persone che giocano abitualmente al Superenalotto possano, per una volta, rinunciare al montepremi per ricostituirlo la volta Come ho detto, ci affidiamo a lei e al Governo, perché è un'idea che va tutta costruita e verificata, ma credo che l'obiettivo e l'intento siano chiari. Senatrice Adamo, ci faremo carico di trasmettere al Governo domattina questa vostra proposta, consapevoli della delicatezza del momento che sta vivendo il Paese

voti).* Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1503, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.